influenza il sistema dell'economia del Paese, perché l'emittenza locale ha una diretta connessione con le produzioni locali.

teniamo, e facendo affidamento anche sul corso dei lavori parlamentari (cioè sul completamento dell'esame del disegno di legge finanziaria presso l'altro ramo del Parlamento),

il Governo ad assumere ogni opportuna iniziativa volta a prevedere, nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria, un incremento degli incentivi

con stanziamenti pari a 70 milioni di euro per l'anno 2010, 90 milioni di euro per l'anno 2011 e 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Per chiarezza di esposizione, si tratta di risorse già previste dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, che aveva destinato alle emittenti locali una cifra pari a 250 milioni di euro,

Credo che questo sia un ordine del giorno importante e che potrebbe essere anche sottoscritto, in perfetto stile *bipartisan*, da tutti i colleghi presenti in Aula quest'oggi. Spiego il perché: non esiste un senatore o un deputato che nella sua vita politica non abbia rilasciato una dichiarazione o un'intervista a una radio o a una televisione locale. Quindi tutti quanti noi conosciamo perfettamente il ruolo essenziale svolto in questi trent'anni dall'emittenza locale televisiva e radiofonica: si tratta di un servizio pubblico che spesso si è trovato a dover supplire alle carenze del vero servizio pubblico offerto dalla concessionaria pubblica, cioè la RAI. pubblica, cioè la RAI. Tutti quanti noi conosciamo perfettamente il significato e il valore dell'attività di queste centinaia di emittenti locali televisive e radiofoniche che operano sul territorio, offrendo lavoro a giornalisti, operatori e pubblicitari e creando un indotto straordinario anche per la nostra economia e per le piccole e medie imprese. So che possiamo contare sulla sensibilità del Governo, come ci è stato ricordato dal vice ministro Vegas e da altri colleghi che abbiamo contattato e con i quali abbiamo lavorato per la soluzione di questo problema. Sarà proprio la sensibilità del Governo a far sì che questo

gli incrementi e gli incentivi previsti dalla legge, saranno decine e decine, per non dire centinaia, le piccole imprese del mondo radiotelevisivo che saranno costrette a chiudere. concludere l'intervento ringraziando per la sensibilità dimostrata sia il relatore Saia sia i componenti del Governo che qui si sono alternati.

che motivano, con parole che sentiamo da 17 anni, l'opportunità di aderire al contenuto di questi due emendamenti.

Non possiamo chiedere che si voti perché, per prassi consolidata, nel momento in cui i primi firmatari decidono di trasformare un emendamento in ordine del giorno, bisogna parlare di quest'ultimo. Vorrei però far notare, signor Presidente, che identico ordine del giorno è stato approvato dall'Assemblea nel maggio scorso.

(e di fatto con questa scelta rende nulla, qualora non l'avessimo capito, qualsiasi incidenza degli ordini del giorno) o questo è il segno di una nostra sostanziale inutilità.

che vi siano dialogo e capacità di interlocuzione. Però, in questa finanziaria non avete aperto nessuna finestra: vi siete chiusi. E anche davanti ad emendamenti oggettivamente espressione della maggioranza dell'Aula ci troviamo di fronte ad un Governo chiuso, che impone ai senatori della maggioranza di ripiegare

che prevede anche una normale copertura finanziaria (ricordo perfettamente quella legge, che fu fatta proprio per dare spazio reale all'emittenza locale), atteso che siamo ancora in quella situazione veramente ambigua in virtù della quale il servizio pubblico radiotelevisivo è coperto non soltanto dal canone ma anche da abbondante pubblicità, che viene quindi sottratta al mercato della pubblicità delle televisioni locali.

Qui in Senato, d'altronde, i colleghi sanno che ci siamo scontrati con molti problemi di copertura, che hanno impedito la soluzione di diverse questioni. L'impegno è quello di definire il problema al più presto (auspicabilmente,

in riva al mare o sulle sponde dei laghi naturali di maggior rilievo nazionale, e comunque situati in un contesto territoriale a forte valenza turistica, con particolare riguardo ai Comuni già titolari di concessione.

che ci viene rappresentato come problematico, ossia quello delle possibili connessioni con il riciclaggio e con il sistema di infiltrazione della criminalità organizzata, sono contestabili precisa scelta dello Stato di intervenire con una presenza vigile su queste strutture, che costituiscono un'importante integrazione all'offerta turistica di alcuni territori.

a vocazione turistica, al fine di riequilibrare un'offerta che esiste in altra parte del Paese e che oggettivamente, per quanto ci riguarda, è penalizzante.

Signor Presidente, su questo argomento credo di dover esprimere un totale dissenso

il documento da me presentato in Commissione antimafia sul gioco d'azzardo, in generale, e sulle case da gioco, in particolare. Non è questa la strada per risolvere i problemi del turismo italiano né dello sviluppo del Mezzogiorno. Non lo è. Questa è una scorciatoia pericolosa anche rispetto alle iniziative annunciate dal Ministro per il turismo, perché la mafia, la 'ndrangheta e le organizzazioni criminali invece di comprare le case da gioco compreranno gli alberghi a cinque stelle per poter gestire anche questa parte del turismo di qualità. *(Applausi dai Gruppi sono le infrastrutture, i servizi, l'offerta turistica, il *marketing*, l'immagine internazionale del nostro Paese, non le case da gioco.

solo una battuta: di fronte alla mancanza di assunzione di responsabilità da parte del Governo su problemi gravi, mi stupisco, ci stupiamo, siamo scandalizzati - uso volutamente questo termine - che questo termine - che vi prendiate la briga di prevedere nuove case da gioco. Credo che ciò sia immorale verso quei cittadini che si aspettano risposte concrete da questa finanziaria e da questo Governo.

riemerge il tema delle case da gioco. Penso però che il Parlamento si possa fidare dei lavori svolti dalla Commissione parlamentare antimafia nel corso di più legislature, con diverse maggioranze e diverse sensibilità.

che per attrarre investimenti oggi si richiede una condizione fondamentale: tenere lontana la mafia dai territori. Ecco perché il Parlamento,

la risposta del Governo, ed è bene che su questo il Parlamento dia un segnale chiaro all'Europa e al Paese: venite nel Mezzogiorno perché vogliamo attrarre investimenti sani e siamo pronti a tenere lontano la mafia. Al contrario, quella avanzata è una

il relatore e il Governo hanno deciso per l'accantonamento. Oggi si scioglie il nodo dell'accantonamento attraverso

cambiando addirittura all'ultimo secondo la propria posizione, il relatore e il Governo debbano accogliere l'ordine del giorno illustrato dal senatore Baldini. E non vi è ragione perché venga accolto l'ordine del giorno del

comunque per spingere un disegno di legge che, invece, deve essere discusso nella Commissione competente - lo ripeto per la terza volta - nella più ampia libertà. Non possiamo far pensare che da quest'Aula, con tutta la contrarietà che è emersa, sia uscito in qualche modo, attraverso una formulazione anche generica, un ordine del giorno che dimostra comunque la volontà del Parlamento, ma soprattutto la volontà del Governo, di andare avanti sull'istituzione sull'istituzione di nuovi casinò. Quindi, pregherei il relatore e il Governo di rimanere fermi sulla loro posizione (invito al ritiro o parere contrario), revocando la propria disponibilità ad accogliere ordini del giorno di qualsiasi tipo e lasciando che un problema così

Signor Presidente, premesso che in materia di casinò il Parlamento vota ordini del giorno da vent'anni e non se ne sono mai fatti,

manifestata una disponibilità ad accogliere tale ordine del giorno. Tuttavia, registrato l'umore complessivo dell'Assemblea, non ho difficoltà a chiarire meglio il pensiero del Governo relativamente alla questione, preannunciando un parere contrario nel caso in cui venisse presentato un ordine del giorno in materia.

ragionevoli per una parte e condivisibili per l'altra. Per quanto mi riguarda, l'idea di una riflessione più pacata più attenta alle diverse questioni, da sviluppare in Commissione attraverso un disegno di legge organico, mi pare metodologicamente corretta. Se però l'umore è quello che l'Aula ha manifestato rumoreggiando, se questo

che il Parlamento decida per l'eliminazione del gioco d'azzardo nella forma dei casinò ed è legittimo che lo Stato provveda invece a recuperare importanti risorse attraverso una implementazione delle lotterie nazionali, che anch'esse producono danni importanti per le famiglie. Lì però vi è una ragione alta, nobile, ossia l'implementazione delle entrate per lo Stato. Quello che non è accettabile è il pregiudizio per cui ciò che è possibile al Nord non può essere fatto al Sud. Ho chiesto in modo provocatorio, parlando anche con qualche tecnico della materia concernente la sicurezza pubblica, se sia possibile istituire case da gioco ove il controllo rigorosissimo dei flussi fosse garantito attraverso un livello di accertamento elevatissimo.

chiara cognizione che è possibile ipotizzare l'istituzione di case da gioco in condizioni di tranquillità in merito al riciclaggio. Ma il tema dell'indotto a cui si riferisce il senatore Lauro è oggettivamente inquietante: quell'indotto non può valere soltanto per le aree del Sud, perché Saint Vincent, Venezia, Campione o Sanremo non sono realtà diverse per quanto riguarda i processi di tipo speculativo e per quanto riguarda non solo il riciclaggio, ma anche l'usura. Allora, il Governo vada in Commissione con una proposta. Mi va benissimo che sia quella dell'abolizione. Signor Presidente, intendo porre due ordini di problemi.

coloro che rappresentano nel Parlamento, e qui in Senato, questi Comuni hanno tutto l'interesse a bloccare qualunque iniziativa che miri ad aumentare il numero delle case da gioco perché, come si suol dire, Credo che la difesa fatta da parlamentari che hanno interessi specifici nelle città di provenienza in cui esistono i casinò sia una posizione scontata che, in quanto tale, ha poca rilevanza sul piano strettamente politico della valutazione complessiva del problema.

da quando sono parlamentare - cambiare in un senso e nell'altro il proprio parere. La storia parlamentare è piena di migliaia di casi in cui il Governo, di qualunque maggioranza sia stato espressione, ha, nel corso dell'*iter* dei lavori parlamentari, cambiato la propria posizione.

Signor Presidente, ribadisco l'importanza di arrivare a una soluzione del problema dei crediti che le aziende vantano nei confronti della pubblica amministrazione. Ne abbiamo parlato con il Vice Ministro. Credo che tale questione sia importante anche per le Regioni, perché nel momento in cui c'è una compensazione dei debiti tra imprese ed enti locali, riusciamo a far emergere

è opportuno mantenere molto rigidi i cordoni della borsa in un momento in cui anche, da ultimo, l'Unione europea ha raccomandato una intensificazione dell'azione di rientro di tutti i Paesi europei, appunto perché in una fase di difficoltà economica è opportuno mantenere mantenere salda la linea della finanza pubblica. Quindi, anche su iniziative che sarebbero di per sé interessanti e che saranno perseguite dal Governo (probabilmente non subito, ma nel prossimo futuro e auspicabilmente nell'arco della legislatura),

di valutazione comparativa tra i diversi livelli di imposte, nella consapevolezza che una diminuzione della pressione tributaria è indispensabile per assicurare qualche possibilità di sviluppo al Paese allorquando uscirà della crisi. Forse occorre fare una sorta di menù

la cosiddetta cedolare secca sugli affitti (misura che sarebbe estremamente ragionevole) va vista in un quadro comparato. Poi, ovviamente, vi è un problema di copertura. senatore Baldassarri sono molto interessanti, ma in qualche caso comporterebbero alcuni problemi di funzionamento dell'amministrazione. Sotto questo profilo, questo profilo, quindi, il ragionamento di diminuzione della pressione fiscale, pur assolutamente condiviso dal Governo, deve essere affrontato non immediatamente in questa fase ma, come io spero, già dal prossimo anno, quando saranno più chiari i canali

tutto il Parlamento e consentire di risolvere finalmente quel problema del "tassa e spendi" che ci ha portato nelle condizioni economiche e finanziarie in cui ci troviamo oggi.

Premetto che l'intero pacchetto di emendamenti non scioglie nessun cordone della borsa: nessuno di questi emendamenti determina aumenti di deficit pubblico, in quanto ciascuno di essi è totalmente coperto da tagli di spesa.

alla voce degli acquisti di tutte le pubbliche amministrazioni, può essere nel tempo problematico il taglio nella dimensione che ci siamo permessi di indicare, che è semplicemente la correzione di quella gobba di esplosione di spesa avvenuta negli ultimi cinque o sei anni. credo che i cittadini italiani che hanno dovuto subire l'aumento di tasse a fronte di quell'aumento di spesa possano esprimere un giudizio positivo in termini di maggiore maggiore quantità e migliore qualità dei servizi sociali ottenuti. Diverso è invece il ragionamento sull'altra voce di spesa, quella

dal giorno dopo e, quindi, tali da poter consentire una certa copertura dei provvedimenti contenuti in questi emendamenti. La ragione

Quindi, non si tratta di mollare i cordoni della borsa, bensì di assumere la responsabilità di incidere su quei due bubboni di spesa pubblica che hanno spesso determinato elementi di connivenza tra economia, politica e organizzazioni criminali. Mi rendo conto che il processo è lungo e difficile e che va affrontato con una grande compattezza della politica e delle istituzioni, sia della maggioranza, sia del Governo, sia dell'opposizione. È un percorso lungo che richiede determinazione, e ha ragione il vice ministro Vegas a dire che non si fa con la bacchetta magica. Tuttavia, se non si comincia mai, se non si comincia mai, è evidente che chi beneficia di queste acque torbide ha l'assicurazione che mai si arriverà all'obiettivo.

ma è il ragionamento accorato di chi guarda ai bisogni delle famiglie, delle imprese, del tessuto sociale ed economico del nostro Paese e sa non si potrà ridurre quella oppressione fiscale se non riducendo la spesa pubblica corrente. Non è che rinviando a tre o a cinque anni anni potremo ridurre la pressione fiscale aumentando il deficit: non lo si può fare oggi e non lo si potrà fare mai! Quindi, chi assume la responsabilità di ridurre il peso opprimente (per i tartassati, non per gli evasori) del fisco, sa che assume la responsabilità di aggredire con tagli strutturali e permanenti quelle voci di spesa.

ed assumono entità rilevanti. Ma non si può modificare con la politica economica l'andamento tendenziale inerziale se non con una manovra quantitativamente rilevante: man mano che riduciamo le quantità dell'intervento riduciamo le possibilità potenziali di incidere su quegli andamenti tendenziali. Nonostante questo, mi rendo conto e prendo atto della posizione espressa dal vice ministro Vegas. Quindi, per quanto riguarda gli 3.0.3 e 3.0.5, accetto l'invito a presentare un ordine del giorno,

ed i fondi per la ricerca scientifica e tecnologica, accetto l'invito al ritiro, presentando un ordine del giorno che indichi nelle possibili entrate dello scudo fiscale, di carattere *una tantum*,la possibilità di procedere a finanziare tali interventi, che sono altrettanto *una tantum*. Questo per sgombrare il campo da ogni equivoco. Le entrate che deriveranno dello scudo fiscale, essendo *una tantum*, non hanno nulla, ma nulla a che vedere con provvedimenti strutturali e permanenti. sarebbe in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione. Restano infine, signor Presidente, tre emendamenti.

il collega Garavaglia ha già illustrato ieri il contenuto. Esso non presenta alcun problema di copertura. La discussione avvenuta tra noi e i colleghi della Lega era proprio sulla forma di copertura; la Lega proponeva

di 6 miliardi di euro di fondi perduti in credito di imposta, coprendo il credito di imposta per il valore di 2 miliardi Tutti sanno che 6 meno 2 fa 4, quindi 4 miliardi di euro di risorse che così si liberano andrebbero a finanziare l'esclusione dei salari dalla base imponibile dell'IRAP per tutte le piccole e medie imprese al di sotto di 50 addetti, mentre per tutte le imprese al di sopra di 50 addetti tale esclusione avverrebbe *pro quota* rispetto al totale degli occupati dell'azienda. Questo è l'emendamento, che non tocca alcun euro delle entrate delle Regioni, perché, come ha già detto il collega Garavaglia, la formula che proponiamo è è quella della detrazione dalle altre imposte dirette ed indirette; quindi, le Regioni ricevono l'IRAP per intero e l'azienda porta questa quota a detrazione delle imposte dirette e indirette.

l'inizio del percorso degli sgravi IRPEF per la famiglia. Nell'emendamento originario è da una parte, il taglio di 15 miliardi di euro nella voce "acquisti" e, dall'altra, la concessione di deduzioni per carichi familiari di 5.000 euro all'anno, per un equivalente di 15 miliardi. Questo permetterebbe una doppia progressività dell'IRPEF, verticale in base al reddito e orizzontale a parità di reddito, in base alle teste che sono da sfamare dentro lo stesso nucleo familiare. tale riformulazione, fermo restando il taglio di 15 miliardi che potrà essere realizzato nel tempo, si propone di partire con una deduzione di 1.000 euro soltanto per ogni componente del nucleo familiare. Quindi, potenzialmente si tagliano 15 miliardi di euro ma si propone di usare adesso soltanto 3 miliardi, per avviare tale percorso. Peraltro, così riformulato l'emendamento non farebbe altro che rendere strutturale e permanente il provvedimento assunto lodevolmente ieri dal Governo. Nel momento in cui il Governo ha ridotto l'acconto IRPEF per 3,8 miliardi

quindi, non modifica la pressione fiscale, ma è positivo. C'è da aspettarsi qualche elemento che però non riduce la positività dell'intervento, perché tutti sappiamo che il giudizio dei mercati finanziari,

di alcuni Soloni editorialisti, che confondono la cassa con la competenza, la riduzione dell'acconto semmai determina quest'anno un fabbisogno di cassa favorevole a tutto questo. Così riformulato, l'emendamento non fa altro che rendere parzialmente strutturale e permanente in termini di competenza largamente coperta quanto il Governo ha deciso ieri in termini di cassa.

e il taglio di 2 miliardi per coprire quell'*escamotage* puramente tecnico del primo anno di scopertura; si può partire, allora, con una deduzione sugli affitti di 1.000 euro soltanto per il primo anno. Questo riduce l'onere tecnico-ragionieristico a 500 milioni per il primo anno,

Forse è bene informare i colleghi del contenuto dell'emendamento 3.0.4

la richiesta di porre in votazione i tre emendamenti che ho illustrato in precedenza.

3.0.9 (testo 2) contiene soluzioni in tema di trattamento fiscale degli affitti assolutamente identiche, o in ogni caso assai simili, a quelle quelle previste nell'emendamento 3.0.800, di cui è prima firmataria la presidente del Gruppo del Partito Democratico,

Signor Presidente, posso capire le ragioni per le quali gli emendamenti precedenti hanno avuto il parere contrario del Governo e del relatore,

quali siano le ragioni di equilibrio finanziario che spingono il relatore ed il Governo a dare parere contrario sull'emendamento 3.0.9 (testo 2) e su quello assai simile, il 3.0.800, del Partito Democratico. La La scelta si spiega solo nel senso di un Governo che vuole restare assolutamente immobile di fronte alla crisi. Abbiamo infatti convenuto, ed il Governo ha dovuto ammettere, che la norma che modifica il trattamento fiscale degli affitti - sia nel senso di introdurre un prelievo ad aliquota unitaria del 20 per cento sull'affitto percepito, sia nel senso di introdurre una deduzione a favore dell'inquilino che paga quell'affitto - certamente nel primo anno produce un onere, che si riduce però significativamente nel secondo, fino ad annullarsi nel terzo. Non è dunque seriamente sostenibile, signor Presidente, signor Vice Ministro,

detrazione significativa o deduzione sull'affitto pagato. La stessa proposta, dunque, nei programmi elettorali, la stessa soluzione negli emendamenti, un dibattito che ha appurato l'equilibrio finanziario di questa proposta e la sua sostenibilità: perché adesso non dire di sì? Posso capire per gli altri emendamenti, ma per questo è assolutamente incomprensibile. Per questa ragione, invito i colleghi della maggioranza, di fronte all'emendamento 3.0.9 (testo 2) del senatore Baldassarri, a modificare il loro orientamento: colleghi, se voterete a favore, non farete altro che attuare il programma di Governo sulla base del quale avete ottenuto la fiducia di un così grande numero di elettori

Senato: giornate e giornate di discussione e la passione di tanti colleghi senatori che avanzano proposte di modificazione legislativa che si traducono in nulla,

sono inviti al Governo perché esamini l'eventualità di adottare, forse, qualche provvedimento. Su questa materia, come ha detto testé il collega Morando, è veramente possibile determinare una convergenza con l'opposizione? Sono firmatario di un disegno di legge su questa materia, che è agli atti del Senato, per l'introduzione della cedolare secca.

Abbiamo vissuto nel nostro Paese alcune esperienze, come quella delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, stimate all'inizio dalla Ragioneria dello Stato come impraticabili perché comportanti oneri attraverso la rinuncia al gettito, al gettito, ma rivelatesi poi positive sia dal punto di vista del fisco - perché hanno permesso l'emersione dal nero di importanti comparti dell'edilizia - sia in generale per l'economia, perché hanno riattivato un settore fondamentale. La misura della cedolare secca sugli affitti produce esattamente, anche se non in un tempo immediato, questo risultato: riattiva risorse per l'economia, muove il patrimonio abitativo soprattutto a vantaggio delle giovani coppie, di chi vuole accedere alla casa,

conclusiva della legge finanziaria, nella quale molto si è discusso e nulla è stato approvato, affinché qualcosa con questa votazione possa essere approvato. *(Applausi

e dei circa 60 subemendamenti ad essi riferiti. Esaurita la fase delle votazioni degli emendamenti sul disegno di legge finanziaria, si passerà alle votazioni degli articoli 2 e 3, alle dichiarazioni congiunte di voto finale sui disegni di legge finanziaria e di bilancio, nonché alla votazione finale del disegno di legge finanziaria con scrutinio nominale elettronico. La seduta sarà quindi sospesa per consentire al Governo di presentare la Nota di variazioni al bilancio e alla 5a Commissione di esaminarla e presentare le proprie conclusioni all'Assemblea. Una volta definiti tali adempimenti, la seduta riprenderà per la discussione e votazione della Nota di variazioni, nonché per la votazione finale con scrutinio nominale elettronico del disegno di legge di bilancio. **Interrogazioni, annunzio**